sono in corso gli accertamenti del perché questo è accaduto: ci sono delle commissioni che stanno lavorando. In merito all'evento fornisco gli elementi di dettaglio ad oggi in mio possesso, che naturalmente sono soggetti a cambiamenti e modifiche, man mano che gli accertamenti saranno fatti. Come noto, il giorno 24 luglio, verso le ore 4 del mattino, nella stazione di Roma Tiburtina è scoppiato un incendio che ha causato la completa distruzione dell'apparato di sicurezza CEI, un apparato centrale elettrico ad itinerari, destinato alla gestione e al controllo della circolazione dei treni. L'incendio ha interessato i locali tecnologici, ed in particolare la sala relè, ubicata in parte al piano seminterrato, al piano terra ed al primo piano del fabbricato viaggiatori. Allo stato degli accertamenti, sulla base di notizie ricevute dalle Ferrovie dello Stato, possiamo oggi fornire i seguenti primi dati, che il personale addetto alla circolazione treni presente nella sala di comando degli apparati di Roma Tiburtina notava verso le ore 4 del mattino la presenza di fumo nei locali di propria pertinenza e attivava prontamente le procedure previste dal piano di emergenza della cabina. Secondo; in particolare, venivano allertati gli organi esterni addetti alla gestione dell'emergenza incendio (Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco), oltre ai dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Oltre ai Vigili del fuoco, interveniva sul posto il personale del Gruppo come previsto dal piano di emergenza, che prestava tutta la propria collaborazione richiesta dai Vigili del fuoco, e in particolare la messa in sicurezza degli impianti elettrici attraverso il sezionamento delle sorgenti di alimentazione. Inoltre, allo stato attuale, sono in corso i necessari accertamenti circa le cause dell'incendio. A tale scopo, oltre alle indagini avviate dalla magistratura e dalla commissione d'inchiesta istituita da Rete ferroviaria italiana, ho istituito una commissione d'indagine ministeriale, composta da tecnici del Ministero e dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che fornirà le conclusioni in tempi rapidi: in 60 giorni dovranno farmele pervenire. La commissione ministeriale è già stata convocata presso la stazione Tiburtina per un primo sopralluogo nell'area interessata. Non appena saranno concluse le attività d'inchiesta sarà ovviamente possibile verificare le cause che hanno generato il rogo e, quindi, anche eventuali responsabilità. Sulla sicurezza del cantiere e il piano di emergenza, faccio notare che il fabbricato interessato dall'incendio si trova al di fuori dell'area di cantiere per i lavori di *restyling* e di potenziamento della stazione. In merito alle preoccupazioni sulla sicurezza dei cantieri, sempre le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che tali lavori, di particolare complessità, sono stati affidati ad imprese dotate di elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano l'operatività dei cantieri temporanei e mobili. In particolare, tali disposizioni prevedono adeguate attività di vigilanza da parte dei soggetti a ciò individuati dalla normativa di legge. In merito ai piani di emergenza, mi è stato precisato che, ai sensi delle norme vigenti, occorre, in esito alla valutazione dei rischi di incendio, adottare le necessarie misure organizzative e gestionali riportandole in appositi piani di emergenza redatti secondo precisi criteri. A seguito di una mia richiesta, sono stato informato che la stazione di Roma Tiburtina ha, in attuazione di tali norme, redatto il piano nel 2005 e lo ha aggiornato nel 2010. In particolare, è stato predisposto, informando tra gli altri il competente Comando dei Vigili del fuoco, apposito piano di emergenza interno della cabina di Roma Tiburtina. Ritengo però opportuno ribadire che, prima di avere certezze in merito al corretto funzionamento del piano di emergenza, dovremo

delle Ferrovie dello Stato ha informato il mio Dicastero che, per quanto concerne il ripristino del servizio ferroviario, già nella giornata di domenica 24 luglio sono stati riattivati i collegamenti da Roma a Firenze e viceversa, garantendo nella stessa giornata di domenica circa il 60 per cento dell'offerta a lunga percorrenza programmata e il 50 per cento dell'offerta metropolitana sulla tratta Fiumicino-Orte. La tratta metropolitana Tiburtina-Tivoli è stata deviata sulla stazione di Roma Termini, garantendo circa il 75 per cento dell'offerta, e sono stati predisposti servizi di navetta sostitutivi. Nei giorni successivi si è provveduto a consolidare i provvedimenti infrastrutturali e di esercizio delle prime ore, consentendo il recupero della gestione delle infrastrutture necessarie a garantire l'offerta commerciale sulle linee interessanti la stazione di Roma Tiburtina, riuscendo così a garantire nella giornata di lunedì 25 luglio l'80 per cento dell'offerta a lunga percorrenza, portandola al 90 per cento nel giorno successivo sulle tre direttrici che si diramano dalla stazione Tiburtina, compresa quella prevalentemente interessata dal traffico pendolare. Per quanto riguarda l'offerta regionale, sulla tratta Fiumicino-Orte, quella maggiormente interessata dai pendolari e dai viaggiatori che si recano presso l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, di Fiumicino, informo che, a fronte di una diminuzione dei treni circolanti, è stata raddoppiata la composizione del materiale rotabile, in modo da garantire circa l'80 dei posti offerti rispetto al programma previsto prima dell'evento, e dal 26 luglio è stata ripristinata la fermata per il servizio viaggiatori alla stazione Tiburtina. Ad oggi i treni circolano, ma ovviamente si registrano ritardi, soprattutto sulle tratte regionali. Sulla lunga percorrenza e Alta velocità, Trenitalia ha avviato il 27 luglio la piena offerta estiva; il numero di corse di tale offerta, in vigore fino alla fine di agosto, sarà tuttavia potenziato per tutto questo fine settimana con sette Frecce Alta velocità aggiuntive al giorno. Dal 26 luglio, poi, la stazione di Roma Tiburtina è tornata agibile con entrambi gli ingressi, lato Pietralata e lato Nomentano, ed è stata riaperta la fermata Tiburtina della linea B della metropolitana. Per quanto attiene all'assistenza alla clientela, da domenica sono stati molti gli operatori straordinari messi in campo dall'impresa ferroviaria e sono stati già disposti rimborsi di biglietti, per un valore complessivo di circa 680.000 euro. di Trenitalia 800892021 sono state attivate circa 100 postazioni fisse, il 50 per il numero delle chiamate è comunque in rilevante calo rispetto ai primi giorni. Infine, per quanto Ferrovie dello Stato stanno predisponendo un programma di riattivazione completa degli impianti di controllo e comando del traffico ferroviario completamente distrutti dall'incendio, in vista anche della massiccia affluenza di viaggiatori previsti per i primi giorni di agosto. Per quanto attiene il ripristino completo degli impianti dell'apparato centrale della stazione Tiburtina, è stata avviata, anche alla luce del nuovo ruolo che si accinge ad avere lo scalo in questione, la progettazione per l'installazione di un più moderno apparato centrale computerizzato, analogamente a quello già realizzato nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense, Roma San Pietro e Roma Smistamento. In conclusione, l'incendio presso la stazione Tiburtina di Roma ha determinato una situazione molto seria e di non facile gestione. Mi sembra però che, grazie all'impegno profuso a più livelli di responsabilità, l'emergenza sia stata gestita in modo apprezzabile,

I nostri sforzi saranno tutti orientati non solo a scoprire le reali cause del rogo ma anche ad evitare, ovviamente, che simili accadimenti si possano ripetere. Voglio dire al Presidente e ai colleghi senatori che naturalmente, man mano che mi perverranno notizie

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, apprezziamo come ogni volta la sua sensibilità e disponibilità; ci dispiace però constatare che la relazione che le è stata preparata è stata purtroppo, a nostro avviso, insoddisfacente e sicuramente insufficiente. A distanza di quattro giorni dall'accaduto, il Governo non è ancora in grado di formulare una serie di ipotesi circostanziate, suffragate e attendibili, e devo dirle sinceramente che in questo contesto è apparsa davvero insopportabile la sensazione mediatica di scaricabarile che abbiamo avvertito e continuiamo ad avvertire a diverse riprese e da diversi soggetti, in ultimo anche da autorevoli esponenti del suo Dicastero. Prima i No TAV, poi il furto di rame dei rom, da cui lei - devo dargliene atto - ragionevolmente ha preso una qualche distanza, oggi l'ACEA e il sindaco Alemanno, con scambio di accuse e minacce reciproche. Di questo passo, c'è da aspettarsi, nell'attesa degli accertamenti, che si possa anche assistere ad indagini nei confronti degli ebrei, degli omosessuali e magari anche dei comunisti, che fanno sempre notizia.

grazie

Come lei sa - ne abbiamo discusso qualche settimana fa proprio in quest'Aula e, con mozioni approvate da tutto il Senato - è stato chiesto di essere messi a conoscenza di questi fondamentali documenti Ministro, ancora non abbiamo, nonostante le reiterate e formali richieste, anche da parte della Commissione competente. Se incontriamo così tanta fatica per avere documenti dovuti, che peraltro un Governo che opera con trasparenza dovrebbe rendere pubblici, proprio per fugare i dubbi di discrezionalità e arbitrii nell'organizzare i servizi pubblici, non oso supporre le difficoltà che incontreremo per farci raccontare le possibili cause e i conseguenti responsabili.

verrebbe da dire, tanto più fragili quanto più gli apparati si sono specializzati e sono stati innovati per essere più sicuri. Inoltre, il tema dei costi di esercizio è risultato essere più delicato degli investimenti per gli impianti da realizzare. È evidente che qualcosa alla base non funziona, e a poco vale riproporre le mille domande che ci siamo fatti fatti in questi giorni, dalle segnalazioni d'allarme alle cause attendibili del guasto, al sistema dei soccorsi e di pronto intervento (che proprio pronto, a dire il vero, non è sembrato), al ripristino delle condizioni normali di esercizio.

Credo che così facendo, negli anni l'Italia sia stata ridotta a un Paese non in più grado di affrontare tempestivamente non solo le calamità, ma anche le semplici nevicate, il maltempo e da ultimo anche gli incendi. I guasti colposi o dolosi non avvertono né per telefono né, purtroppo, in tempo. Ministro, siamo però d'accordo con lei: nessuno è attrezzato per i miracoli, ma per evitare disastri bisognerebbe dar prova di effettiva volontà di volerli scongiurare; inoltre, quando purtroppo avvengono, capire come mai si sono verificati e renderne conto è semplicemente doveroso.

Signor Ministro, l'incidente occorso nella stazione di Roma Tiburtina offre oggi lo spunto per accendere ulteriormente i riflettori sullo storico problema dell'inaccettabile inadeguatezza infrastrutturale del nostro sistema dei trasporti su rotaia,

Lo stesso Libro bianco 2001 dell'Unione europea sui trasporti imponeva la crescita e il miglioramento del trasporto ferroviario a servizio delle persone e delle merci anche al Sud, non solo con l'importante obiettivo di minimizzare gli inquinamenti ambientali generati nell'ecosistema dai trasporti, ma soprattutto nella consapevolezza che la marginalità geografica, propria soprattutto delle isole, si può eliminare progressivamente grazie ad una sana politica di interventi di miglioramento e riqualificazione del sistema della mobilità, favorendo anche l'intermodalità e la logistica.

Se l'Unione europea abbandona questa linea non è perché il destino è cinico e baro o vi sia una cattiva volontà di quel sistema di governo, ma perché l'attuale Governo mostra disattenzione e disimpegno rispetto a quest'area territoriale. In una fase di crisi economica e finanziaria, quando le risorse scarseggiano, è chiaro che anche l'Unione impegna i propri fondi sui progetti ritenuti più importanti e meglio sostenuti politicamente.

il dottor Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Pare sia essenziale per la vita della Repubblica e per le comunicazioni del nostro Paese. Quando vi fu

Credo che una volta per tutte si debba stabilire che questo dottor Moretti si occupi di altre attività, magari agrituristiche o gastronomiche, e lasci in pace le Ferrovie dello Stato.

il destino sovrasta il dottor Moretti. Non comprendiamo però perché il dottor Moretti debba sovrastare la felicità dei passeggeri delle Ferrovie dello Stato.

Signor Presidente, signor Ministro, pur apprezzando la cortesia e la celerità con la qual è venuto in Senato a riferire le informazioni in suo possesso,

Castelli), riparte con polemiche ed insinuazioni: veniamo così a scoprire che non c'era l'acqua

che il tempo di 60 giorni, di fronte ad un comportamento così stravagante, ai limiti dell'irresponsabilità, di autorevoli membri del Governo, sia un tempo biblico, enormemente lungo.

insinua l'idea che dietro queste cose ci sia un'azione combinata che mette insieme pezzi delle istituzioni e altro, è evidente che si rischia di far degenerare ulteriormente

i disagi hanno riguardato soprattutto le tratte regionali (anche se è la verità) senza affrontare il nodo di un equilibrio tra la gestione regionale di parte della rete e la gestione nazionale.

una delle opere più moderne in Italia, per poi scoprila così vulnerabile poche ore dopo. Di fronte a questi temi bisogna poi stabilire quali sono e quali saranno in futuro le priorità, perché la sensazione è che questo problema

abbiamo ascoltato con attenzione la ricostruzione della dinamica degli eventi accaduti domenica 24 luglio e degli sforzi fatti per ripristinare una situazione di normalità.

che sul tema della sicurezza e dei controlli in Italia vi sono ancora molte zone d'ombra, che necessitano di essere rimosse immediatamente. Vi sono responsabilità tecniche ed amministrative che dobbiamo lasciare alla commissione d'inchiesta che lei, signor Ministro, ha prontamente formato e di cui le diamo atto. Vi sono anche responsabilità penali (se ed in quanto ci sono), delle quali se ne deve occupare la magistratura e vogliamo che solo essa se ne occupi. Ciò detto, affermo che non permetteremo che il livello della sicurezza nel nostro Paese possa venir meno, che vigileremo affinché la verità venga appurata e i responsabili siano individuati. Siamo stufi, però, del balletto delle attribuzioni di colpe e responsabilità, come abbiamo avvertito anche su questa vicenda, in maniera più o meno esplicita (dal sindaco Alemanno al vice ministro Castelli). Ciò che ci interessa davvero non è soltanto la dinamica dell'evento, ma è anche capire una volta per tutte i rischi potenziali cui il nostro Paese è inconsapevolmente esposto ogni giorno, ignaro ignaro degli effettivi standard di sicurezza e controlli applicati. Parliamoci chiaramente: domenica scorsa l'incendio è accaduto alla stazione Tiburtina, in un quartiere densamente popolato, dove le abitazioni distano solo poche centinaia di metri dalla palazzina che è andata completamente in fiamme. Ministro, i residenti della zona, d'ora in poi, a sentirsi sicuri, a non aver paura che un giorno o l'altro i sistemi di monitoraggio delle centraline elettriche non funzionino?

Probabilmente si dovrebbero riconsiderare le enormi spese per il rifacimento della stazione, in gran parte dedicate a spazi commerciali e al nuovo nodo dell'alta velocità, alla luce della necessità di più adeguati investimenti per garantire una reale sicurezza di sistema. Siamo convinti che ogni scelta di investimento e miglioramento delle infrastrutture di trasporto debba essere fatta solo dopo aver garantito per le strutture in uso la massima sicurezza possibile, per viaggiatori e lavoratori. lei ieri ha detto di essere scettico sull'ipotesi che a provocare il corto circuito possano essere stati i prelevamenti di cavi elettrici da cui ricavare rame. Eppure, al di là del fatto che il rogo sia imputabile o meno al furto, ricorderà che numerosi erano stati i campanelli di allarme al riguardo negli ultimi tempi. In Italia i furti di questo metallo sono in costante aumento, come denunciano le statistiche delle forze dell'ordine. Tra l'altro, mentre mentre Tiburtina era in fiamme, la TAV Roma-Firenze era già ferma di suo, perché a bloccare l'alta velocità ci aveva già pensato un furto di cavi a Settebagni, alle porte della capitale. A giugno, sulla ferrovia Roma-Ostia, si è registrato il *record* di 3 furti in una sola settimana. Non crede che anche questo costituisca un problema di sicurezza da affrontare quanto prima? E poi la notizia data dall'associazione Codici, che ha denunciato l'assenza di controlli nei cantieri della stazione. Una condizione di totale mancanza di sicurezza. La sicurezza, signor Ministro, è una condizione che non si raggiunge una volta per tutte, ma va migliorata giorno dopo giorno. Occorre una programmazione continua e sistematica negli investimenti nella rete, negli impianti e nelle infrastrutture. C'è bisogno di formazione continua di tutti gli addetti ai lavori, di procedere sistematicamente a manutenzione e controlli delle apparecchiature.

Non posso tralasciare il fatto che gli eventi verificatisi chiamano pesantemente in causa il sistema di *governance* del settore dei trasporti. C'è stata una gestione disastrosa sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai viaggiatori, lasciati soli nel caos più totale. Da lungo tempo ormai il Gruppo Italia dei Valori si è impegnato a denunciare i disagi subiti dai cittadini che scelgono il trasporto su ferro. Ma lei, Ministro, si è dimostrato avviso - poco attento ad ogni forma di segnalazione. Anche in questa occasione, a seguito dei primi disagi, dopo le polemiche sollevate dai passeggeri dei treni pendolari, lei ha richiamato gli italiani ad un «maggiore senso di responsabilità». Ha detto loro che nessuno è attrezzato per i miracoli. Signor Ministro, non si possono proferire parole del genere, secondo la nostra opinione. E' capitato a tutti, più volte, di leggere negli esercizi pubblici cartelli dal tono ironico con scritto: «per i miracoli ci stiamo attrezzando». Ebbene, lei si è spinto oltre, dicendo che non siete attrezzati. Non dovrei essere io a ricordarle che lei è membro del Governo e che il Paese pretende un Governo che si assuma per intero le responsabilità. Abbiamo apprezzato la disponibilità e la prontezza nel venire subito a riferire in Parlamento, aspetti che non sfuggono, ma che riteniamo non un atto straordinario, bensì un atto dovuto. Ma, la prego, non continui a fare dichiarazioni di questo tipo. Sono un insulto ai cittadini. E poi, sarebbe meglio

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la gravità dell'evento impone di tenersi lontani da ogni possibile strumentalizzazione o contrapposizione faziosa. L'incidente ha colpito il primo scalo di nuova generazione dell'alta velocità ferroviaria, poco prima della sua inaugurazione, con ripercussioni sull'intera mobilità metropolitana romana e sull'intera rete ferroviaria italiana. Ringrazio il Ministro per essere venuto ad

bisogna fare una constatazione sulla vulnerabilità della nostra rete. In un Paese come il nostro, dove esiste una pianificazione trasportistica e logistica molto ampia, talvolta sovrabbondante, ci rendiamo conto delle ripercussioni logistiche, economiche, sociali, persino strategiche, derivanti da fatto che il Paese possa restare tagliato in due per molte ore, per qualche giorno, e con disagi di qualche settimana? pensate delle misure per ridurre la vulnerabilità del sistema in relazione alla entrata in crisi di un singolo nodo? Una riflessione ben più urgente riguarda il problema del monitoraggio e del controllo. È stata distrutta la sala operativa di una stazione fra le più importanti d'Italia, vitale per la mobilità di tutto il Paese. È possibile che non ci fossero, o non funzionassero, i più normali e banali allarmi antincendio e antifumo? Funzionavano? C'erano? Erano previsti o dovuti? Lo stesso per i rilevatori «Le misure antincendio a Tiburtina sono insufficienti» avevano denunciato i ferrovieri, nero su bianco, sulla rivista «Ancora in marcia». E le stesse Ferrovie dello Stato hanno ammesso in un comunicato che non c'è stato dal sistema alcun avviso di quanto stava accadendo. Il fumo è stato notato a vista, e per caso, da alcuni addetti gli operatori di polizia privata, addetti al presidio della stazione nelle ore notturne, che stavano facendo? Quanti sono, e come operano? Chi ne organizza l'operatività? Ci sono state anche polemiche sulla facilità di accesso al cantiere: il 18 luglio, una settimana prima, alcuni associati di un comitato di cittadini hanno dimostrato, con tanto di foto,

un po' troppe. Sicuramente, è stata decisiva la scoperta tardiva, di cui abbiamo appena detto, e, secondo alcune fonti, anche la difficoltà di accosto dei veicoli del Vigili del fuoco (e questo sarebbe grave). È stato certamente decisivo - lo ha detto ufficialmente il capo ufficio stampa dei Vigili del fuoco - il fatto che quel giorno fosse sospesa l'erogazione dell'acqua in quella parte di Roma. E le autobotti con cui si domano gli incendi nelle foreste? Ma soprattutto, secondo un comunicato ufficiale dell'ACEA, «la rete idrica al servizio della stazione Tiburtina è sempre rimasta alimentata secondo le normali condizioni di fornitura, con particolare riferimento alla rete antincendio; infatti per tale zona non era previsto alcun disservizio, né si è verificato». Questo il comunicato ufficiale dell'ACEA. Secondo altri, i Vigili del fuoco sono intervenuti subito, e lo hanno visto tutti, ma non in forze: solo con due veicoli. Per altro verso, sembrerebbe che i Vigili del fuoco abbiano dovuto aspettare che, solo dopo molte ore, i responsabili di RFI disattivassero la corrente ad alta tensione nei settori andati a fuoco. terzo ordine di riflessioni riguarda le cause e le responsabilità. Qui i palleggi di responsabilità sono anche di più. L'incendio è avvenuto all'interno dell'area di cantiere delle Ferrovie dello Stato, e si è sviluppato all'interno della cabina elettrica. Qui le domande sono molte: ad esempio, nella cabina elettrica erano in funzione due relè, uno recente e collaudato, l'altro vecchio.

escluse, quindi si lascia intendere che è la terza. Nelle stesse ore, nel campo nomadi di via Salone vengono sequestrati un quintale di cavi di rame che potrebbero, ma anche no (e qui forse si poteva evitare una pericolosa e odiosa speculazione), provenire da Tiburtina. Intanto, però, viene fuori che il furto del rame è una cosa consueta, che tutti conoscono, pur sapendo benissimo, gli addetti ai lavori, che la conseguenza è il sovraccarico delle linee elettriche rimaste e, di conseguenza, il rischio di incendio "anche in tempi differiti". In tempi differiti? Ma vogliamo scherzare? Ciò vuol dire che non c'è neanche il controllo su quanto è stato preventivamente rubato e che, in seguito, può causare incendi. In conclusione, davvero il quadro è molto confuso. Sono passati pochi giorni e quanto ho detto non intende essere una critica al Ministro, che è venuto qui e ha tenuto una relazione con gli elementi che aveva. Io non so francamente dire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno; non vorrei, parafrasando Brecht, che come diciamo di Rembrandt che se fosse nato nato senza mani avrebbe dipinto allo stesso modo, dovessimo dire un giorno di qualche responsabile di questa vicenda che se fosse nato senza testa avrebbe agito allo stesso modo.

e gli sviluppi di questa grave situazione che si è venuta a creare dopo il violento incendio divampato - lo ricordo - solo quattro giorni fa nella sala apparati della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.

e la pericolosità determinata dalla presenza di cavi dell'alta tensione. Ovviamente ai lavoratori e ai volontari che si sono impegnati nell'emergenza deve essere riconosciuta la nostra gratitudine di parlamentari e cittadini.

solo a chi utilizza regolarmente il treno per i propri spostamenti ma anche a chi, in questo periodo estivo, sta utilizzando il trasporto ferroviario per le proprie vacanze. scalo di Roma Tiburtina, infatti, ha costretto i treni a transitare a bassa velocità per l'assenza di segnali elettrici, determinando forti ripercussioni sulla rete ferroviaria dell'intero territorio nazionale. Ritardi di ore si sono avuti nei principali snodi della linea ad alta velocità e delle altre linee, con migliaia di passeggeri costretti ad attese estenuanti sotto le pensiline, a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Napoli.

tratte a rischio di soppressione o ritardi. Probabilmente le risposte a queste domande devono essere fornite in primo luogo da Trenitalia che - ne siamo certi - sta studiando un piano strategico per supportare l'emergenza immediata e anche quella prossima futura. Ci auguriamo Ci auguriamo quindi - chiediamo anche un interessamento a tal proposito al Ministro - che il personale della compagnia ferroviaria sia a disposizione del pubblico per rispondere alle legittime domande sollevate dagli utenti, intensificando anche i servizi di sportello diretto con i cittadini e la presenza di personale all'interno delle stazioni per spiegare in che cosa consistono le restrizioni al traffico ferroviario, di cui parlano tutti i giornali, e i riflessi sui normali servizi ai viaggiatori. La preoccupazione a breve termine riguarda quindi il prossimo mese e i problemi che i residenti e anche i turisti si troveranno ad affrontare, e speriamo sempre con minore difficoltà man mano che passano i giorni. la preoccupazione a lungo termine è sicuramente più grave e riguarda l'intera stazione Tiburtina. Sono in corso da alcuni anni lavori di ristrutturazione per renderla quello che vuole essere, ossia un nodo cruciale per l'alta velocità. Speriamo che questo grave incidente non causi troppi rallentamenti nella prosecuzione dei lavori e che sia presto garantito un servizio di qualità agli utenti. Si parla di un numero importante di circa 22 milioni di utenti all'anno. Roma - Tiburtina è fondamentale per il raccordo con le grandi città del Nord Italia e per garantire un buon livello di efficienza ai treni ad alta velocità che forse, nell'immaginario comune di molti, sono esclusivamente lo strumento che dà modo ai passeggeri più ricchi di viaggiare più rapidamente tra due città,

questo grave incidente possa apportare variazioni sulle tempistiche e sui costi di realizzazione. Per le tempistiche, ricordiamo che, nel 2007, l'allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, aveva assicurato la conclusione entro due anni. Oggi, a distanza di 4 anni da quelle dichiarazioni, non vorremmo fossero trovate altre scuse per ritardare la chiusura del cantiere. Per i costi di realizzazione, il progetto originario prevedeva una galleria sopraelevata di 300 metri, con un investimento di 155 milioni di euro, in parte pubblico e in parte proveniente dagli introiti della trasformazione urbanistica delle aree vicine. Sembra che l'incendio abbia interessato non le parti di nuova realizzazione, ma la vecchia centrale di controllo dei treni: una struttura che aveva circa 20 anni e che non era interessata dai lavori, ma che aveva una grande importanza strategica per il controllo dei mezzi in transito nel Centro-Italia. In conclusione, mi auguro che, dopo i necessari accertamenti per garantire la messa in sicurezza dell'area, riprendano prontamente i lavori, ma presumibilmente i danni economici saranno ingenti e il rischio è che il cantiere romano possa anche fermarsi, speriamo di no. Chiediamo quindi al Ministro di relazionare in quest'Aula, appena avrà a disposizione i dati necessari, sulla quantificazione dei danni subiti dalla stazione e sul reperimento delle risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, nonché sulle tempistiche necessarie alla conclusione del progetto. Aspettiamo quindi il Ministro al più presto per essere messi a conoscenza sull'evoluzione dei fatti, lo ringraziamo e siamo

offrire ai giornalisti una *location* particolare, la nuova stazione ferroviaria, per presentare la sua nuova giunta, e ciò invece è venuto meno perché l'amministratore delegato ha fatto sapere che per motivi di sicurezza ciò non era possibile. La spiegazione

nel Governo della Repubblica alcuni autorevoli rappresentanti non avvertono l'esigenza di mantenere uno stile e una misura che, viceversa, vengono chiesti all'opposizione. Risulta tuttavia preoccupante il fatto che i Vigili del fuoco abbiano stentato ad intervenire con rapidità.

con asprezza sui giornali come la Regione, in modo particolare, abbia tardato ad intervenire. Ciò va anche al di là del colore politico che oggi caratterizza un'amministrazione regionale. il nostro decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nel nuovo testo, ha aperto grandi prospettive, ma se poi queste ultime non vengono organizzate seriamente, si rischia di determinare una serie di controindicazioni.

che riemerge a causa di questo incidente: dobbiamo individuarlo con molta correttezza.

può essere accaduto che non sia scattata alcuna protezione automatica. Bisogna capire, senza per questo sostituirci ai tecnici, a coloro che si intendono di mestiere di queste cose, l'origine di questo incidente, che al momento nessuno è in grado di valutare.

l'apparato più avanzato per regolare questi traffici. La stazione Tiburtina sarà sempre più importante e strategica. Paradossalmente, potremmo dire che se un incendio si fosse verificato a Roma Termini, i disagi sarebbero stati assai minori rispetto

gli uffici delle Ferrovie, l'incidente non produrrà conseguenze in ordine alla tempistica per la inaugurazione della nuova stazione. Questo secondo quanto sostengono gli uffici: poi vedremo cosa

L'amministratore delegato ci ha sempre detto che le Ferrovie italiane sono, a confronto con altre ferrovie, la società che impiega più denaro di altri

non c'è la scelta - il Governo può confermare - di penalizzare il Sud, impedendo che l'Alta velocità da Napoli prosegua per Reggio Calabria, Messina e Palermo. È una divagazione giornalistica pubblicata da «Il Sole 24 Ore»:

Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Palermo. Quindi, quella notizia apparsa sulla stampa, segnatamente su «Il Sole 24 Ore», è un'invenzione giornalistica non suffragata da alcuna

Ritengo pertanto che dobbiamo rimanere in attesa dei risultati delle commissioni, evitare di raccogliere le sollecitazioni che molto spesso i *mass media* fanno le polemiche di cui abbiamo visto protagonisti tanti operatori politici del posto. Capisco che il Sindaco abbia ritenuto di intervenire, chiedendo che i responsabili rispondano di quanto è successo. Tutto bene, però credo che ci dobbiamo

Già guardare e osservare i volti anche dei senatori della stessa maggioranza, ci ha fatto capire che questa fiducia è giunta come un fulmine a ciel sereno, perché assolutamente immotivata. Non c'era assolutamente la necessità d'interrompere una discussione, che sarebbe durata

uno schiaffo che viene dato al Senato e al Parlamento, e dimostra l'arroganza con cui questo Governo procede in questa legislatura, particolarmente in materia di giustizia. Noi abbiamo cominciato la nostra mattinata di lavori in Senato ricordando con le parole del nostro collega Giaretta come la questione finanziaria ed economica richiami la la massima attenzione di tutto il Paese, di tutte le categorie, di tutte le associazioni e sindacati che congiuntamente hanno elevato un grido di protesta e hanno chiesto interventi concordi, decisi e forti nel settore dell'economia. Il Governo ha risposto mettendo la fiducia sul disegno di legge che riguarda "il processo lungo" e che riguarda, ancora una volta, delle norme a tutela innanzitutto del presidente del Consiglio Berlusconi per far saltare i suoi processi. Al di là di questa prima motivazione e di questo schiaffo che con arroganza è stato dato al Parlamento, direi che questa fiducia si pone come un altolà nei confronti di una parte della stessa maggioranza e, in particolare, nei confronti dei senatori della Lega Nord. Ci sono infatti quanto meno due motivi per cui da una parte della maggioranza, e da parte dei senatori della Lega non era assolutamente accettabile un disegno di legge di questo tipo.

vuol dire non rendersi conto della fortissima contraddizione, della negazione di se stessi e della politica che si va facendo sul territorio. C'è inoltre un motivo più specifico e più tecnico, se vogliamo, che forse non è stato nemmeno visto da tanti senatori della maggioranza, contenuto esclusivamente all'interno del maxiemendamento. È il riferimento che è stato fatto all'interno dell'emendamento aggiuntivo

per legare le mani da un punto di vista politico, ma anche tecnico, alla Lega, la quale prepotentemente viene bloccata nelle proprie eventuali intemperanze, contestazioni o, comunque, insoddisfazioni.

è un provvedimento che non può assolutamente essere difeso all'esterno di quest'Aula nemmeno da parte dei membri del Governo e dei senatori della maggioranza. Infatti, ci si è dimenticati

la possibilità di votare sulla politica del Governo sulla giustizia (perché questo era il significato di quel *referendum*) e il popolo italiano ha bocciato decisamente, in maniera netta e senza possibilità di false interpretazioni quello che ha fatto il Governo in questi tre anni in materia di giustizia. È stata una bocciatura completa e ora - peggio che fare orecchie da mercante il Governo, con arroganza e prepotenza, ripropone norme che vanno a tutela innanzitutto del Presidente del Consiglio dei ministri. E come lo fanno? Lo dico in due parole perché ormai è stata ampiamente esaminata tale questione nel corso dei vari interventi che ci sono stati nella giornata di ieri e nel corso di questa mattina. Si interviene modificando il sistema di acquisizione della prova, che era un sistema ben articolato, equilibrato, armonico e rispettoso dell'articolo 111 della Costituzione perché era stato modificato ripetutamente proprio per consentire la pienezza e la regolarità del contraddittorio tra le parti.

dovrà eliminare solo quelle «manifestamente non pertinenti». Qui c'è una giravolta completa che stravolge il sistema di acquisizione della prova. Abbiamo già fatto degli esempi chiarissimi; io stesso avevo fatto riferimento a un delitto che si dovesse verificare in un mercato all'aperto, o addirittura in uno stadio, come quello di San Siro: tutti coloro che sono presenti all'evento delittuoso possono dire cose pertinenti al delitto che si verifica e, se il difensore fa richiesta di sentire e mette in lista-testi 10, 100, 1.000 o 80.000 persone, queste, essendo tutte pertinenti e non essendo, ragionando *a contrariis*, manifestamente non pertinenti

che rivolgo anche a loro. Vorrei sapere se il senatore Mugnai, firmatario dell'emendamento che contestiamo, e il senatore Mazzatorta hanno letto tutto il loro emendamento, perché a mio parere si sono fermati alla prima parte, alla lettura della modifica dell'articolo 190 del codice di procedura penale, e si sono dimenticati di leggere, o comunque di commentare, la modifica dell'articolo 495 del codice di rito penale, cioè quella che riguarda i poteri del tribunale e del giudice. Anche in quel caso, caso, essi vogliono inserire una norma che fa riferimento, ancora una volta, alle prove manifestamente non pertinenti. Quindi, tutta quella specie di arringa, quasi infuocata e degna forse di miglior causa, del senatore Mugnai è assolutamente infondata, perché anche all'articolo 495 - si è dimenticato di dirlo - hanno inserito la questione relativa alle prove manifestamente non pertinenti. Ancora una volta si pone quindi per

questa nullità sappiamo benissimo che, essendo di carattere generale, può essere impugnata fino in fondo, in tutti i vari gradi di giudizio. per chi avesse mai dei dubbi - ma credo che questi non li abbia nessuno, tantomeno i senatori della maggioranza - che è una norma che serviva a tutti i processi personali del presidente Berlusconi.

secondo l'accusa, i prosseneti del presidente Berlusconi. Guardate, mi sono limitato, visto che si parla di *escort* e di testimoni su questa materia, a prendere l'elenco del telefono o a scorrere Internet e ho recuperato centinaia di pagine che riguardano centinaia e centinaia di

norma nuova, con il loro disegno di legge, non potrà assolutamente dir loro di no. Credo allora che questa norma, signor Presidente e signori senatori, produca effetti assolutamente negativi e devastanti, perché è direi proprio di immediata evidenza

nell'ambito dei quali è imputato il presidente Berlusconi: il processo Mills, il processo Ruby e tutti gli altri per violazione di norme finanziarie e valutarie. Le conseguenze di questa portata, soprattutto e purtroppo, non si limiteranno al presidente Berlusconi, ma riguarderanno tanti altri procedimenti per fatti criminali, anche gravi e molto gravi, e questo alla faccia di chi invoca la sicurezza e di chi pretende sul territorio di avere sempre maggior sicurezza e sempre maggiori tutele, e poi in Parlamento fa esattamente il contrario. Questa norma è un passo ulteriore verso quella che sarà la paralisi della giustizia penale, settore che già versa

personalistiche, alla cancellazione delle esigenze di giustizia e di sicurezza. Il cittadino che ci guarda, che ci legge, che sente quello che stiamo facendo in Parlamento Parlamento avrà sicuramente l'idea di un legislatore o di una politica schizofrenica, perché da una parte si dice una cosa, e poi concretamente de ne fa un'altra. Si tratta di una considerazione oggettiva, perché, se da una parte, in questo momento, alla Camera dei deputati si sta cercando di abbreviare i termini della prescrizione, quindi di accorciare sostanzialmente il processo per la rapidità del giudizio, in questa sede stiamo facendo esattamente il contrario; si crea quindi una sinergia

e noi continuiamo a dirvi che di questo passo la giustizia andrà sempre peggio, la macchina della giustizia non avrà alcun miglioramento e sarà destinata veramente a una paralisi. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando ha un contenuto del tutto diverso e stravolto da quello approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio scorso. A conferma di un Governo in stato confusionale e profondamente in crisi, nonostante la nomina del nuovo Ministro della giustizia, arriva puntuale la richiesta dell'ennesima fiducia: altro che il confronto costantemente auspicato dal presidente Napolitano! Dal processo breve siamo passati al processo lungo, ma mi pare che si voglia arrivare ad una sorta di non processo, introducendo il principio per cui la legge non è uguale per tutti. A mio avviso, il disegno di legge in esame avrà l'effetto di stravolgere ancor di più l'*iter* processuale e non garantirà in nulla la certezza della pena. Ancora una volta si ha la percezione netta che questo provvedimento costituisca una norma transitoria a favore del Presidente del Consiglio e che la maggioranza stia facendo di tutto per garantirgli l'impunità. La proposta che viene sottoposta alla nostra attenzione si articola, sostanzialmente, in due punti, colleghi: divieto di ridurre le liste dei testimoni (ma se non viene fissato un limite, i tempi sono destinati ad allungarsi e a diventare biblici) e non utilizzabilità del fatto accertato in un altro procedimento. Scelta pericolosa, questa, che innescherebbe la conseguenza immediata di ridimensionare fortemente l'autonomia del giudice, il quale risulterebbe anche condizionato nelle valutazioni relative ai tempi del processo. La competenza del giudice, insomma, resta limitata alla sola manifesta non pertinenza della prova: un parametro del tutto inadeguato alle esigenze processuali perché sganciato dal merito processuale e dal complessivo contesto probatorio. Il disegno di legge sul processo lungo mette in evidenza l'allungamento dei processi, e noi non possiamo non notare che esso si pone in forte contrasto con i temi del processo breve, all'esame dell'altro ramo del Parlamento e già precedentemente discusso dal Senato. che il processo breve conterrebbe elementi conflittuali con la nostra Costituzione; allo stesso modo e a maggior ragione - mi permetto di sottolineare quello lungo o infinito, che ha inizio e non ha fine (come nell'ambito della geometria descrittiva si definisce una semiretta), incidendo direttamente sull'autonomia e sull'indipendenza del magistrato, sarebbe palesemente incostituzionale. Alla fine, l'allungamento dei tempi si incrocerebbe con l'accorciamento della durata del processo, sino alla prescrizione del primo, artificiosamente. E vorrei chiedere: è eticamente corretto avere una prescrizione da questo punto di vista? Insomma, questo provvedimento andrebbe ad ingenerare ulteriore confusione, infliggendo un *vulnus* all'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancita dalla nostra Costituzione. Nell'avviarmi a concludere, pongo una domanda, cari colleghi e colleghe, che contiene già in sé la risposta: si può prevedere un processo apparentemente lungo fino a quando quello breve non l'avrà spazzato via? Pertanto, cerchiamo tutti insieme di recuperare quel senso dello Stato smarrito da questi "provvedimenti spezzatino", affrontiamo seriamente la riforma della giustizia, al di là degli annunci puntualmente e spudoratamente smentiti. Altro che certezza della pena e giusto processo: così si arriverà a destabilizzare ancor di più le istituzioni, mettendo a repentaglio l'equilibrio sociale e democratico del nostro Paese, già fortemente provato da varie crisi, di cui quella più drammatica è legata al futuro economico di milioni di italiani, che non hanno certezza

insisterò su tre punti. Il primo concerne l'importanza della ritualità delle nostre procedure parlamentari. abbiamo avuto un'interruzione della discussione generale - come ricordava poc'anzi il collega Casson - quando eravamo in pochi a dover ancora intervenire, i tempi erano certi e non c'era alcun bisogno di una forzatura improvvisa. Il ministro Vito è arrivato in Aula leggendo un foglietto e farfugliando parole che a malapena si capivano, dicendo che il Consiglio dei ministri aveva posto la fiducia.

per la dignità di tutto il Parlamento: non solo dei parlamentari dell'opposizione, ma anche di quelli della maggioranza. Tutti teniamo a queste ritualità. Anche il modo in cui la presidente Mauro, subito dopo le parole farfugliate e quasi incomprensibili del ministro Vito, ha immediatamente chiuso la discussione generale non dando neanche il tempo di capire bene le parole del ministro rientra in uno stile di Presidenza non accettabile,

quest'ottica, l'apposizione della questione di fiducia in Parlamento è una cosa seria, un momento solenne in cui in Parlamento il Governo impegna la sua esistenza. Quindi, dovrebbe essere fatta con una ritualità

secondo punto che vorrei sottolineare è che in questi giorni e nelle scorse settimane il neosegretario del Popolo della Libertà Alfano

ha dichiarato di volersi ispirare in particolar modo al popolarismo europeo e all'insegnamento sociale della Chiesa, che potrebbero essere molto utili in questo caso specifico di un voto di fiducia su una legge *ad personam*. Penso che il segretario Alfano, in vista di questa costituente popolare, potrebbe in particolar modo ricordare un documento molto importante della Conferenza episcopale italiana dell'anno 1991, «Educare alla legalità».

(cioè in favore di qualcuno)» in forma di ricatto riducono «drasticamente le leggi «generali», vanificando così le istanze di chi non ha voce né forza. Per le stesse ragioni il Parlamento corre il rischio di essere ridotto a strumento di semplice ratifica di intese realizzate al suo esterno». Voi oggi siete riusciti, con il voto di fiducia su una legge *ad personam,* ad andare platealmente contro questo documento che parla di leggi particolaristiche e di Parlamento ridotto a ratificare. dunque volete davvero ispirarvi a questo pensiero, cercate d'ora in poi di fare il contrario di quello che avete fatto oggi. Più in generale, questo documento si ispira a una classica visione sul ruolo dell'autorità e della legge che merita di essere richiamata. La si può trovare in una ottima citazione di San Tommaso,

«La legge umana in tanto è tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza». La legge di oggi, essendo una legge *ad personam,* rientra perfettamente in questa censura che possiamo far risalire, come visione di fondo, a San Tommaso.

In tale *referendum* quella legge, presa ad esempio tra le leggi *ad personam*, è stata rigettata dalla grande maggioranza del corpo elettorale italiano, compresi gli elettori del centrodestra. È possibile che dopo un verdetto del genere voi sfidiate di nuovo non solo il corpo elettorale italiano, ma anche il vostro elettorato?

richiamare un'altra elezione binaria della storia costituzionale francese, utile, soprattutto, per come si conclude. Siamo nella campagna elettorale del 1877 il *leader* repubblicano Gambetta pronuncia queste parole: «Quando la sola autorità davanti alla quale bisogna che tutti si inchinino si sarà pronunciata, non crediate che qualcuno possa essere in grado di tenerle testa. Non crediate che quando questi milioni di francesi, contadini, operai, borghesi, elettori della libera terra francese, avranno fatto la loro scelta, e precisamente nei termini in cui la domanda è posta, non crediate che quando essi avranno indicato la loro scelta e fatto conoscere la loro volontà, non crediate che, quando tanti milioni di francesi avranno parlato, ci possa essere qualcuno, a qualsiasi livello della gerarchia politica o amministrativa, che possa resistere. Quando la Francia avrà fatto sentire la propria voce sovrana, credetelo bene signori, non si potrà che sottomettersi o dimettersi». Il corpo elettorale vi ha chiesto di sottomettervi al suo verdetto contro le leggi *ad personam.* Non vi volete sottomettere? Vi dovrete presto dimettere. Signor Presidente, in conseguenza dell'emendamento 1.1000 presentato, il titolo del disegno di legge viene così sostituito: «Modifiche agli articoli 190, 238-*bis*, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354».

di legge discusso dall'altro ramo del Parlamento o quello presentato da alcuni colleghi parlamentari. Anche la modifica sostanziale e sostanziosa del titolo che il sottosegretario Caliendo

sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ma ci troviamo di fronte a un altro

del primo atto del nuovo Ministro oppure se è stato il primo atto di cui il vecchio Ministro non ha voluto assumere una sorta di paternità politica o una responsabilità se non altro morale.

ai colleghi parlamentari e alle forze politiche che su un modo di proporsi all'opinione pubblica costruiscono spesso effimere fortune elettorali.

non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente e puntualmente elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua, l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto sia la pena di morte. Non sono parole mie, ma di Aldo Moro, rispetto alle quali immaginavo ci potessero essere una discussione in quest'Aula e un confronto tra le diverse sensibilità. Purtroppo la questione non è più questa. Non parliamo più

appena sono tornati preminenti gli interessi giudiziari del *Premier*. Questo è il motivo per cui ormai questo verrà ricordato come un provvedimento che riguarda esclusivamente il processo lungo. Ancora una volta

dal testo la norma che prevede di ascoltare i testimoni che hanno contribuito a determinare sentenze di condanna passate in giudicato usate come prova. stato pronto a confrontarmi sul fatto che un qualsiasi imputato ha il diritto di scegliersi la propria strategia difensiva e processuale.

(sia quelle che potrebbero essere dettate dal buon senso, sia quelle frutto di forzature evidenti, quando non dettate da malafede) siano solo ed esclusivamente introdotte nel nostro ordinamento nell'interesse di qualche processo che, guarda caso, riguarda sempre il Presidente del Consiglio. Infatti, la storiella del processo lungo e la facoltà di fare interrogare testimoni chiamati dalla difesa senza alcun limite, anche allorquando ci si richiama alle stesse condizioni dell'accusa, è evidente che non convince più nessuno. Anzi, in verità il

cosa significa? Che vedremo magari in diretta televisiva qualche giornalista interrogare, nel processo in cui è imputato, qualcuna delle amiche che aveva invitato alle

È questo che verrà fatto - immagino - durante la diretta televisiva? E tra le pause del processo manderemo in onda anche gli *spot* pubblicitari? Ma insomma, guardate che oltre a questi processi ce ne sono altri. Provate ad immaginare cosa può accadere quando lo stupratore, il capoclan, il capocosca, lo 'ndranghetista, il mafioso guarda negli occhi il testimone durante un dibattimento. C'è un limite a tutto. Non è tutto un film in questo nostro Paese, purtroppo.

si rischia concretamente di rallentare tutti i processi penali in corso, a parte quelli per i quali è chiuso il primo grado. del tentativo di allungare i tempi del dibattimento con il ridurre i termini della prescrizione avrà un effetto oggettivamente dirompente. Proprio l'effetto congiunto deve farci riflettere. sono sincero, e ritengo che questa fiducia sia un chiaro ed ultimo segno di debolezza di questo Governo. Questo è un Governo ormai logorato, che è minoranza nel Paese e nell'opinione pubblica, e che, per eterogenesi dei fini, considerato quanto raccontava fino a poco tempo fa il Presidente del Consiglio, non avendo più il consenso nel Paese e nell'opinione pubblica, essendo condannato anche dagli stessi sondaggi sempre sventolati in ogni trasmissione televisiva, sta in piedi solo grazie a quel teatrino della politica, che trova qualche teatrante anche nelle Aule parlamentari e che consegna, in maniera sbagliata e offensiva per il Paese, una maggioranza solo parlamentare. Non avete più la maggioranza nel Paese e io credo che sia opportuno che valutiate seriamente, (altro che fiducia), la possibilità che vi dimettiate.

sull'emendamento presentato dal Governo su cui è stata posta la questione di fiducia. Qualche rilievo tecnico noi dobbiamo farlo, perché questo emendamento presentato dal Governo contiene dei gravi errori, non politici, ma giuridici.

troppo evidenti. Cominciamo dal comma 8 dell'emendamento che interviene modificando l'ordinamento penitenziario. Si dice, alla lettera *a)*, che «i condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-*bis*,

Si viene a creare un mostro, nel momento in cui si collega la morte del sequestrato a un reato che non riguarda il sequestro. Infatti, riguardano il sequestro

Se non consegue la morte, la pena non può essere inferiore a 15 anni. Ora, non si riesce a capire perché, per l'articolo 422, nell'ipotesi in cui vi sia una pena non inferiore a 15 anni, si debba applicare questa esclusione dei benefici penitenziari, mentre per i sequestri di persona a scopo di estorsione o con finalità di terrorismo questo si debba fare, ossia l'esclusione dei benefici penitenziari, solo se c'è la morte. Non si riesce a capire, e chiaramente è un errore, un manifesto errore. La norma è scritta male.

Quanto poi all'articolo 495, si dice che esiste sempre la possibilità per i giudici di escludere le prove superflue.

Ciò significa che, per poterle escludere, devono ricorrere due condizioni: il fatto che siano superflue e manifestamente non pertinenti. Ricorrendone una sola, non si possono escludere. Non ci voleva la congiunzione "e" ma "o", perché radicalmente diversa è la soluzione. Poi ovviamente rimane

1985, le difese furono costrette a chiedere la lettura integrale degli atti al maxiprocesso. Ve lo ricordate? All'epoca Cosa nostra - lo sapemmo dopo - impose agli avvocati di fare quella richiesta. Si trattava di leggere un milione di pagine.

farà un processo nullo, in quanto la sanzione prevista è la nullità. In sostanza, se dei 1.000 testi proposti uno solo non viene sentito il processo è nullo. Ma vi rendete conto di ciò che state introducendo, della devastazione del processo, che da queste norme viene stravolto nel cuore, ossia nell'ammissione dello strumento di prova? Inoltre, a me è dispiaciuto molto sentire ieri il senatore Mugnai dire: ma leggetevi gli articoli, onorevoli colleghi! Chi ha detto che non c'è il filtro non ha letto il codice. C'è l'articolo 468 e il giudice ha il potere di eliminare le liste sovrabbondanti. Guardate, i codici bisogna leggerli, ma bisogna pure capirli.

di mantenere nel nostro codice penale la pena dell'ergastolo. Sarebbe stato un momento anche elevato di dibattito in quest'Aula parlamentare. Ha ancora senso mantenere l'ergastolo? Costituzionalmente

In realtà, il dibattito è decisamente andato in un'altra direzione e anche plasticamente e esteticamente si sta riproducendo in maniera schizofrenica il bicameralismo perfetto così, mentre noi parliamo del processo lungo, nell'altro ramo parlamentare si parla del processo breve.

della necessità di riformare la giustizia italiana. Stamattina vi è stato un importante intervento del Presidente della Repubblica, che ha ricordato lo stato attuale, definendo una «questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile» l'emergenza giustizia nelle carceri. Egli ha parlato di come alla fine si produca «una giustizia deviata», «ritardata e negata»

giudiziari. Ebbene, in quella Commissione, i Gruppi parlamentari, i relatori di maggioranza e di opposizione, il Presidente hanno mostrato che le istituzioni possono ancora dare una buona prova di sé. Si può passare dalle parole ai fatti, si possono prendere provvedimenti per i cittadini, anche per quei cittadini «matti» chiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari, se si vede davvero quando è lesa la dignità delle persone, quando non c'è più il diritto alla salute, quando si va davvero sopra quelli che sono i principi costituzionali, se

Queste parole, nei limiti temporali che mi sono stati dati, sono dedicate a chiedere con sincera franchezza a lei, Sottosegretario, e a lei, collega Mugnai, che ha avuto l'onore della cronaca in questi giorni per un suo emendamento sul processo lungo, perché tutto questo. Quale è la vera

a farsi benedire qualsiasi giustizia giusta, come qualche volta si evoca nei convegni. Inoltre, l'espediente dei testi - non c'è bisogno che lo dica io, bastano quei telefilm di tanti anni fa che ci hanno ammonito su cosa sia l'utilizzo dei testi l'utilizzo dei testi - serve per protrarre in modo indefinito e indefinibile il tempo. Il tempo, collega Mugnai, è una variabile sacrosanta, come ci hanno insegnato i grandi maestri. Non si scherza mai con il tempo. Si possono avere cattive sorprese. il tempo lungo significa che chi si può permettere un buon avvocato o uno studio legale di qualche rilievo non avrà mai la sentenza, e la prescrizione arriverà. Dunque, attraverso questo testo si un doppio risultato: per un verso, la tutela degli interessi di pochissimi, com'è noto, di un gruppo ristrettissimo, uno e poco più di uno, come si sa e come le cronache c'insegnano; dall'altro, si cancella l'opportunità di avere una giustizia corretta per tanta parte della società italiana che invece vorrebbe un processo corretto, un tempo adeguato, delle norme comprensibili. questa legislatura sarà ricordata per le leggi *ad personam* che con questo ultimo articolato raggiungono persino una sorta di epifania. Siamo davvero alla manifestazione più plateale di questo tratto di un Governo che ci auguriamo tutti cada al più presto. (*Segue* VITA). In conclusione, Presidente, la questione è seria e vorrei tanto che anche il rappresentante del Governo, le colleghe ed i colleghi dell'attuale maggioranza ci riflettessero. questa riflessione - di quel percorso transitorio che Antonio Gramsci chiamò crisi di egemonia. È evidente che questo Governo non produce più nessuna egemonia

un fenomeno perverso nelle società democratiche, che non sono più democratiche e che quindi diventano autoritarie e populiste insieme: in tal modo, sfuggono a qualsiasi regola che invece dovrebbe presiedere ad uno Stato di diritto. Non so se tutto questo possa stare a cuore o stia nella testa di chi ha supposto di immaginare questo percorso normativo. rappresentanti del Governo e colleghi, che questo testo non dovrebbe nemmeno esistere. Sembra un incubo. Naturalmente all'atto della fiducia ci sarà questa volta un no molto vivo, anche simbolicamente. Però voglio dirvi: provate a pensarci; guardatevi allo specchio;

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che andiamo ad approvare o, auspicabilmente, a bocciare sulla base di una votazione di fiducia non dovrebbe essere essere trattato nella veste e nella forma in cui viene purtroppo trattato perché, come già abbiamo avuto occasione di ricordare ieri, vi è un articolo del Regolamento del Senato che dichiara inammissibili gli emendamenti estranei estranei all'oggetto del disegno di legge in discussione. Come già abbiamo detto ieri, mi pare assolutamente incontrovertibile che l'ammissibilità dei testimoni in ogni procedimento non abbia nulla a che vedere con l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Tuttavia, anche volendo prescindere da questa premessa, che è pure importante e che testimonia la grave scorrettezza con cui questa maggioranza e questo Governo intendono procedere, credo che oggetto di riflessione debba essere la fiducia che ci apprestiamo a votare. La fiducia è, a mio avviso, un atto inutile e grave che strozza quel dibattito che proprio ieri il presidente Schifani aveva garantito. quindi, si impone in modo del tutto illegittimo e arbitrario sul Parlamento. Il presidente Schifani ha preso un impegno di fronte a tutta l'Aula e il giorno dopo è costretto a rinnegare quell'impegno perché dalla Presidenza del Consiglio gli arriva un *diktat*: far votare la fiducia e impedire un libero dibattito su una riforma che si presenta molto diversa da quella su cui, peraltro, la Conferenza dei Capigruppo aveva all'unanimità disposto un certo calendario. Sappiamo, infatti, perfettamente che la Conferenza dei Capigruppo non era a conoscenza di quel famoso emendamento che travolge l'intero disegno di legge. Quello che è ancora più grave rispetto a tutto questo, che è già di per sé politicamente assai grave, ritengo sia questo modo di fare le riforme su un tema così delicato come quello della giustizia, senza cioè un disegno strategico. Soltanto governicchi fanno cose di questo tipo e piccole e povere maggioranze si apprestano a votare riforme del senza un disegno strategico e inserendo, per altri scopi, emendamenti utili solo ad interessi particolari, ad interessi personali e cioè non utili all'interesse generale del Paese, ma funzionali soltanto a difendere personaggi eccellenti che si trovano coinvolti in procedimenti attualmente pendenti. Ogni riferimento al processo Mills credo che sia del tutto superfluo. Detto questo e, quindi, constatata la totale inadeguatezza di un modo di legiferare che rischia di danneggiare l'impalcatura stessa del nostro sistema giustizia, non posso esimermi anche dal considerare che questa norma sull'ammissibilità dei testimoni, che riduce pesantemente i poteri del giudice,

chiedere di escutere più testimoni possibili per allungare il brodo, per evitare che si arrivi a sentenza e per fare scattare i termini delle prescrizioni. allora, cari colleghi, che una norma di questo tipo mette a rischio il valore stesso giustizia, mette in grave difficoltà quelle parti che si aspettano giustizia dallo Stato, soprattutto, le vittime, le parti lese, quelle che invece vorrebbero che i processi fossero rapidi per ottenere una sentenza che possa riconoscere i propri diritti. Si è detto che questa norma attuerebbe l'articolo 111, comma 3, della Costituzione, che prevede la parità fra difesa e accusa, ma già oggi vi è parità perché il pubblico ministero deve ovviamente soggiacere al giudizio del giudice, il quale può ammettere o restringere la lista dei testimoni proposti sia dal pubblico ministero, che dall'imputato. Semmai il pubblico ministero ha l'onere della prova quindi la sua posizione è ancora più difficile oggi rispetto a quella dell'imputato, di cui si presume la non colpevolezza. Ma credo che, al di là di ciò, vi sia poi anche un principio generale di ragionevolezza delle norme. Questa norma è palesemente irragionevole perché è destinata ad allungare i processi, da qui la denominazione «processo lungo», quando invece

Con una norma di questo tipo, che in sostanza limita di molto la possibilità del giudice di restringere la lista dei testi, si rimette la durata processuale nelle mani della difesa. Voglio citarvi una piccola chicca, un fatto storico che sta a testimoniare come vi sia malafede nelle posizioni del Governo e della maggioranza, perché la strumentalità di tale norma risulta evidente da ciò che accadde un po' di tempo fa. Nel processo Previti la difesa chiese di sentire tutti i magistrati del distretto di Roma, e questo ovviamente per un motivo di facile comprensibilità, cioè per far sì che i tempi scorressero e si arrivasse rapidamente alla prescrizione.

allora come, in realtà, questa norma è stata dettata dagli avvocati del*Premier*, che già in passato in qualche modo avevano cercato di utilizzarla.

riduce la possibilità di utilizzare le sentenze passate in giudicato, nel senso che si consente comunque e sempre alla parte di assumere

il rischio è di allungare ulteriormente la durata dei processi, mettendo in discussione ciò che dovrebbe essere invece già dato per scontato, essendo a fondamento di una sentenza di condanna passata in giudicato. giudicato. Credo che di fronte a tutto questo, cari colleghi, chi ha senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni dovrebbe far prevalere la dignità rispetto alla convenienza personale, dovrebbe far prevalere uno scatto di legittimo orgoglio. Chi ha coraggio dovrebbe in questo frangente storico trovarlo e dire: «Metto a rischio anche la mia candidatura, so che magari il *Premier* si arrabbierà e magari mi depennerà dalla lista dei prossimi candidati per la prossima legislatura, ma credo che la propria dignità personale valga ben più di una ricandidatura». L'interesse generale del Paese ad avere una giustizia che funzioni, che non si concentri sempre e soltanto su norme a difesa di interessi particolare (nel caso di specie gli interessi

Quindi, noi di FLI e di ApI voteremo senz'altro un no convinto alla fiducia, perché vogliamo bocciare questo provvedimento che danneggia la giustizia italiana e molti milioni di cittadini.

pochi ma cari colleghi presenti in Aula, vorrei che i riflettori del Paese inquadrassero l'Aula in questo momento e in queste ore.

e, con una schizofrenia determinata, continuata e aberrante, non finite di farlo.

dei tanti provvedimenti che dal 1994 fino ai nostri giorni sono stati presi. Berlusconi e questa maggioranza hanno ritenuto, senza alcun ritegno, di anteporre le ragioni personali agli interessi del Paese.

lo ripetiamo - va a vergogna del senso civile del nostro Paese, che una volta era considerato la culla del diritto, ma oggi, come

del lessico della lingua italiana. Depenalizzazione del falso in bilancio; mandato di cattura europeo; rogatorie internazionali; introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato (lodo Schifani); legge Cirami sul legittimo sospetto; riduzione della prescrizione, la (si è vergognato pure lui); lodo Alfano, legittimo impedimento e, *in itinere,* intercettazioni telefoniche; lodo Alfano costituzionalizzato; processo breve o prescrizione breve (come ricordavo); ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori: per capirci, la Convenzione di Lanzarote serviva in pratica per ridurre le sanzioni per i delitti commessi con atti sessuali con minori e similari. Camera e Senato della Repubblica sono costati, Berlusconi, il Governo e la maggioranza sono costati al Paese

delle ore d'Aula e Commissione, per cui sappiamo che abbiamo lavorato su questi temi per 731 giorni

ma questo è. Sono i conti della serva, i vostri conti perché questo significa sequestrare il Parlamento, come ho detto nei giorni scorsi. diventa perfino seccante ricordarlo - di conflitto tra politica e magistratura o tra magistratura e politica, è perché di fronte ad una guerra dichiarata dai politici unilateralmente, e i magistrati devono subire l'assalto perché facendo il loro dovere, cercano di applicare la legge in maniera uguale per tutti, politici o meno. Leggevo nei giorni scorsi una bella metafora: visto lo sfascio della giustizia italiana, allungare i tempi indeterminabili del processo è come abbattere una diga mentre incombe un rischio inondazione.

l'ardire, l'impudenza di presentare una norma scritta male che peggiorerà la situazione e farà deragliare completamente il vagone giustizia? Una mela avvelenata che il ministro, o ex ministro, Alfano ha dato al nuovo ministro Nitto Palma il quale,

Scusate, ma si vuole imposturare o continuare a imposturare, come diceva l'aria del Barbiere di Siviglia: ma noi non siamo in un'opera buffa, siamo in Parlamento e voi dovreste governare Questo provvedimento, caro collega Li Gotti, dice due cose. Berlusconi potrebbe essere condannato per due processi: uno è il processo Ruby,

pochissimi ma obbedienti colleghi della maggioranza - come è possibile che non vi rendiate conto che ci troviamo di fronte ad un macigno nella vita della democrazia italiana che va rimosso, e al più presto, perché così ringrazieranno mafiosi, delinquenti,

il voto di fiducia fatelo cadere il Governo! È interesse vostro, per la nostra comune dignità e - se consentite - per la vostra coscienza.

non vorrei e non saprei entrare nel merito tecnico della questione come hanno fatto benissimo gli avvocati, i magistrati ed i costituzionalisti che oggi siedono in questa Aula. Io sono un economista, non sono un tecnico del diritto; sono il lettore di media intelligenza evocato nel suo intervento dal senatore Vita, esattamente come i cittadini italiani. Diciamo pure, nel mio caso, di medio-bassa intelligenza. La differenza è che io ho letto le carte, come è mio preciso dovere i cittadini italiani non lo hanno fatto, come è loro preciso diritto visto che in un sistema democratico delegano la rappresentanza dei loro interessi a delle persone retribuite per farlo, che dovrebbero essere di loro fiducia. Ebbene, il lettore di media intelligenza, o di medio-bassa intelligenza, quale io sono, persino da ignorante del diritto si rende conto di quanto sia assurda una norma che permette quasi a chiunque, purché in grado di pagare un ottimo avvocato, di arrivare alla prescrizione del processo intentato contro di lui attraverso una tecnica dilatoria assurda, consistente nel chiamare a testimoniare soggetti il cui contributo al dibattimento sia anche palesemente irrilevante senza alcun limite di numero mentre, nel frattempo, corre il limite temporale della prescrizione,

ad esaminare una norma che, come questa, danneggia la giustizia italiana e che ha un nome beffardamente opposto rispetto a questa, ribattezzata processo lungo, mentre quella era stata ribattezzata processo breve. Entrambe fanno strage della giustizia italiana: l'una facendo estinguere alcune decine di migliaia di processi (40.000, secondo le stime più ottimistiche) questa rendendo impossibile un numero imprecisato di processi futuri. Ebbene (non se ne ricorderà nessuno, ma io sì) , in occasione del dibattito sul processo breve per la prima volta mi dissociai dal mio Gruppo, che allora era il Popolo della Libertà e adottai un comportamento in dissenso. Allora, in un'Aula piena e tesa parlai di un'agenda nascosta del Presidente del Consiglio dietro l'obiettivo dichiarato di rendere, con quella norma, più brevi i processi che oggi si vogliono rendere lunghi. Oggi no; oggi non parlerò di un'agenda che nella mia ingenuità definivo nascosta perché oggi non è più nascosta per nessuno: è sotto gli occhi di tutti gli italiani ed è un'agenda che mi riempie di un disagio profondo, diciamo pure di vergogna. Avete presente quando ci si vergogna per gli altri? Ecco, io mi sto vergognando per altri e un pochino anche per me stesso. Mi vergogno di vedere approvate queste leggi, oltretutto con il ricorso al voto di fiducia. Allora mi dissociai, con qualche problema di coscienza; non votai quella norma per problemi di coscienza, ma ebbi problemi di coscienza anche a dissociarmi, perché ero comunque perfettamente consapevole che con questo orrendo sistema ero stato nominato, anziché eletto. Per la verità, fui nominato proprio con una scelta *ad personam* fatta dal Presidente del Consiglio, che era il maggiore interessato a quella legge e che mi volle capolista del Popolo della Libertà per la regione Liguria. Ma un conto è la riconoscenza, altro la rappresentanza; e per quanto possa essere stato nominato da un leader, io rappresento e ho continuato a rappresentare i cittadini, per non fare del mio leader il mio padrone. Allora, credo che molti cittadini che alle ultime elezioni hanno votato per

Se aspettavate un'occasione, un momento in cui poter dare voi stessi il segnale di un cambiamento che è nelle cose, che è nel Paese e che spero sia ancora nei vostri cuori, ebbene il momento è arrivato, l'occasione è questa: coglierla dipende solo da voi.

probabilmente stiamo consumando, parlando di giustizia, una battaglia che ha tutt'altro sapore e tutt'altri obiettivi. è buono per dare la famosa spallata. probabilmente ogni strumento è buono per raggiungere l'obiettivo. Si può arrivare alla menzogna, alla maramalderia; abbiamo sentito di tutto ed i veleni si sono sprecati. che la responsabilità di ogni atto di governo è dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene. Capisco che la sinistra sia esperta la storia - ma che oggi si pretenda anche di mettere in atto la dittatura delle opposizioni sembra

Oggi si parla di prerogative relative alla difesa: parliamo di

Sarebbe difficile catalogare un provvedimento che tratta di immigrazione come una legge *ad personam*, che va a toccare gli interessi del Presidente del Consiglio.

Tanto qui uno può dire ciò che vuole e nessuno lo interrompe. Non so se parla per le televisioni o per i pochi che lo stanno ascoltando, ma può dire tutte le sciocchezze che vuole.

se Bersani critica una stampa che per la prima volta muta indirizzo e contesta chi in questo momento cade nelle maglie della giustizia rivendicando addirittura una *class action* contro i giornali perché hanno buttato fango contro il Partito Democratico,

cosa: chi compie un delitto per cui in corso di dibattimento si arriva ad una sentenza che prevede la pena dell'ergastolo, pur anche avendo chiesto un rito abbreviato, non potrà avvantaggiarsi dello sconto di pena connesso alla scelta del rito. Mi sembra talmente pacifico che su questo nessuno ha discusso. È accaduto che nel ragionamento venga attaccato un vagone che non era allacciato originariamente. Al riguardo, suggerirei

Chi ha reminiscenze di studi giuridici ricorda quanto i professori insistevano sul diritto alla difesa, tanto che tutto il codice è permeato attorno al sacrosanto principio del diritto

Questa è filosofia e storia del diritto; la sostanza è: meglio un colpevole libero che un innocente incarcerato. Oggi parliamo esattamente di questo, del diritto alla difesa, del contraddittorio e del fatto che una persona non possa essere condannata per delle prove assunte in un altro processo, dove l'imputato non era presente e non ha potuto chiedere un controinterrogatorio e non ha potuto beneficiare del contraddittorio. Il fatto è dimostrato in un altro dibattimento e compare in un'altra sentenza e l'imputato non ha neanche avuto il modo di controprovare, a sua discolpa.

all'ammissibilità di un teste che possa provare a propria discolpa qualcosa. Oggi, e se ne è parlato a dismisura, il giudice ammette un teste sul criterio della rilevanza. rilevanza. Ma il criterio della rilevanza, pur essendo legge e presente nel codice, è uno dei concetti più sbagliati. La rilevanza avverrà

accompagnatoria. «Si stabilisce la possibilità di esaminare le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione di una sentenza. Questo costituisce un'ulteriore garanzia, per ogni parte processuale, che il verdetto scaturisca dal più ampio quadro istruttorio possibile e non solo da deduzioni logico-giuridiche provenienti da una pronuncia afferente ad altri soggetti».

Voi pensate, conducendo questa battaglia (e se la fate vuol dire che ci credete), che agli italiani non piacciano le leggi *ad personam*. Noi crediamo, invece, che agli italiani non piacciano soprattutto gli speculatori.

mi avrebbe reso più facile l'intervento o, meglio, più specifico e più incisivo. Non è soltanto per avere l'ultima parola, cosa che non mi ha mai affascinato, ma mi sarebbe piaciuto parlare dopo di lui. Al collega Divina devo soltanto dire che ha parlato ignorando la legge, ignorando il sistema processuale. E io temo che abbia parlato come un leghista che abbia paura di scivolare su un terreno politico che la Lega ha sempre combattuto, o ha detto sempre di voler combattere. Il discorso di Divina è significativo, da questo punto di vista. È come se si volesse far credere a qualcuno che loro non hanno capito cosa sia questa legge. È possibile? Ma io non ci credo, perché abbiamo a che fare con dei colleghi intelligenti, e certamente non del tutto ignoranti (parlo del diritto). A me dispiace veramente e sinceramente se qualcuno di voi, o se molti di voi, hanno avuto fastidi allo stomaco. Anzi, dico che è un fattore positivo, perché vuol dire che avete ancora una capacità di reazione, di disturbarvi, ma non per i nostri attacchi, per i nostri tentativi di spallata, che non ci sono stati affatto. Abbiamo tentato di impedire giuridicamente corretto questo termine e politicamente doveroso - che una legge nefasta e negativa come questa possa essere varata e messa nel novero del sistema giuridico italiano, che non la merita. Non è possibile venire in quest'Aula e parlare d'altro, dicendo che la sinistra attacca, specula, dice cosacce e poi nominare Tedesco, Penati. Non c'entra nulla! Questa è una legge vergognosa, l'ennesima legge che avete imposto, anzi state per imporre - per essere più precisi - consapevoli che serve solo al *Premier*! *Premier*! Se venite a dire che pensate che possa servire al diritto alla difesa, devo dirvi con molta sincerità che mi sembra che non abbiate capito nulla della legge, perché essa non ha nulla a che fare con il diritto alla difesa, nulla! Siete partiti bene. Avete ipotizzato di non riconoscere più nel nostro sistema una sensibile riduzione di pena per determinati tipi di reato. L'istituto del rito abbreviato è stato usato ed abusato davanti a certi tipi di reato l'opinione pubblica non accetta questa riduzione, che è sentita come ingiusta. Quindi, era giusto proporre quanto avete proposto, come l'ho proposto io con il mio partito. Eravamo d'accordo, convergevamo. Quando abbiamo opposto resistenza Non c'entra nulla quello di cui stiamo parlando con il diritto alla difesa che è sacrosanto

erra! È già stato spiegato che non c'entra niente il suo richiamo giuridico: questa legge darà la possibilità a tutti i criminali

Questa è la gravità, cari colleghi della maggioranza! Questa è la gravità che stato ignorando, facendovi venire qualche mal di stomaco o allontanandovi dall'Aula, oppure facendo finta o non volendo capire che cosa state per votare. Vi è stato chiesto per gli interessi del *Premier*, perché c'è un processo che vuole far prescrivere, di accettare una legge e di vararla, una legge che è un obbrobrio, che non serve a nulla. al diritto alla difesa, quanti testimoni? Quando mai la difesa di Berlusconi o di altri potenti del momento ha lamentato che i giudici italiani abbiano impedito o impediscano l'acquisizione dei mezzi di prova? Non mi risulta che si sia verificato mai un fatto del genere. Allora non c'era bisogno di dire che si assumono prove a dismisura. Che c'entra il diritto alla difesa con il dire

Poi, perché mettere in discussione le sentenze passate in giudicato? Perché vanificare il lavoro fatto nei processi davanti a tribunali della Repubblica, davanti a magistrati che danno ampie garanzie, per lo meno di trasparenza e di professionalità? Lasciamo stare i casi patologici: perseguiamoli e facciamolo insieme! Facciamo le riforme che non avete voluto fare per rendere la giustizia più funzionante e più trasparente e il magistrato più professionale e più responsabile. Questo vi stiamo chiedendo, e non da ieri.

Non parlo di noi, avvezzi semmai a contrastare le situazioni drammatiche e pericolose, ma di tanti cittadini inermi che dovranno sentirsi interrogare in dibattimento dal *boss*, dal rapinatore, dallo stupratore, dal criminale, dall'uomo potente, direttamente, in quel momento. A chi serviva? A cosa serve introdurre nel processo una tecnica di questo genere? Spiegatelo. Io non posso accettare, sia pure in un'Aula vuota, che mi si venga a parlare della sinistra cattiva e della destra che ha il mal di pancia. Parliamo d'altro. Perché ancora una volta state varando una legge che serve solo a salvare il vostro Capo di Governo, il vostro capo di partito, che tra non molto scomparirà dallo scenario politico, perché questa è la storia? Perché vi state rendendo responsabili? Questo è il punto politico su cui insisto, facendo riferimento a tutti voi, gente con una storia, con una cultura, con una dignità, che varate queste leggi inutili, dannose per il nostro Paese, che non servono a nulla se non agli interessi di una persona. Ecco perché, caro collega Divina, mai come in questo caso l'espressione "legge *ad personam*" è perfetta. È una legge che serve solo ad una persona. Non servirà a nessuno, se non a danneggiare il già difficile cammino e funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Non posso terminare, come ho sempre fatto nei miei interventi, dicendo auspico, penso, spero, esorto, perché so che direi cose stupide. Sono certo, infatti, che voi voterete compatti per mantenere questa posizione e questa maggioranza anche di fronte allo sfacelo che si sta operando nel nostro Paese. ho dovuto dirvelo, perché credo che almeno qualcuno potrà leggere qual è veramente la posizione del Partito Democratico e di queste opposizioni. Abbiamo svolto

*(PdL)*. Signora Presidente, lo scopo del processo penale, lo scopo più avvertito, quello che ha costituito l'insegnamento di tutti coloro che nel processo penale si sono dovuti cimentare, in qualunque ruolo, senatore Maritati, è quello dell'accertamento della verità. Va accertata la verità. Bisogna creare le condizioni migliori perché si possano individuare i profili che consentono una sentenza giusta, ed è in questa direzione, onorevoli colleghi, che bisogna muoversi quando ci si occupa di queste materie. Tutti voi sapete che il codice di procedura penale impone che la prova si costituisca al dibattimento. Il giudice terzo acquisisce gli elementi che gli vengono proposti dall'accusa e dalla difesa, li valuta e quindi assume e quindi assume le sue decisioni. Egli non ha alcuna cognizione, quando il processo comincia, di quali saranno le ipotesi che gli verranno prospettate dalle parti processuali. Davanti a sé ha il capo di imputazione, dove in maniera laconica ed essenziale sono sintetizzate le condotte che formeranno oggetto della sua decisione. Il dibattimento è quella fase dinamica, durante la quale tutto ciò che è utile alle ragioni dei contendenti, delle parti processuali, viene rassegnato al giudice terzo, equilibrato, equidistante, perché egli possa valutare e decidere, stabilire cioè la verità processuale. Trovo francamente bizzarro, signora Presidente, singolare, che argomenti che consentano di sottoporre al giudice una messe più consistente di temi di decisione, di argomenti da esaminare, debbano essere considerati con questa criticità dagli illustri e valorosissimi colleghi della minoranza. La norma non dice che senza alcun criterio si possono segnalare ipotesi al giudice perché le valuti. La norma che ci apprestiamo a votare, e che voteremo con piena convinzione di fare cosa buona e giusta e di dare un contributo affinché l'accertamento della verità, fine ultimo del processo, possa meglio realizzarsi, individua nella manifesta pertinenza le condizioni perché gli elementi di prova possano essere rassegnati al giudice e, qualora questa manifesta pertinenza venisse meno, esistono gli strumenti processuali perché il giudice non accolga le proposte. La reiterazione della pertinenza o degli argomenti pertinenti, la reiterazione di argomenti che sotto ogni profilo valutino la vicenda processuale è un elemento disdicevole? Me lo chiedo, e lo chiedo a tutti coloro che enfaticamente si sono affannati a sostenere che 1.000, 2.000, 3.000 testimoni saranno indotti a tutelare le ragioni esclusivamente di ricchi imputati. La pertinenza è un concetto fondamentale, è un concetto che certamente prevale sulla superfluità, talvolta, anche se, intervenuta l'acquisizione piena delle ragioni che si vogliono introdurre attraverso l'escussione di una serie di testimoni, il giudice, sentite le parti, può disporre che le liste testimoniali vengano sensibilmente ridotte. Francamente, non trovo alcunché di scandaloso in tutto questo, e mi sorprendo dei toni enfatici che sono stati utilizzati per dire che tutto ciò è criminale, che tutto ciò significa la vanificazione di sforzi processuali, che il processo non trarrebbe giovamento da tutto questo, che pochi e noti imputati soltanto ne sarebbero beneficiari. Mi sorprendo, ma uso l'espressione come figura retorica: mi sorprendo senza sorprendermi. Mi sorprendo senza sorprendermi perché questo è il gioco delle parti, perché così si fa, perché se fosse stato altro il contesto nel quale avessimo discusso di questo argomento, i forbiti giuristi che oggi e su questo tema comunque sono intervenuti avrebbero forse proposto soluzioni apprezzabili che avrebbero indotto opportune riflessioni, ma avrebbero compreso e contribuito a che attraverso anche il loro lavoro questo strumento, che consente una cognizione maggiore e più ampia di tutti gli aspetti del processo, potesse diventare legge dello Stato. Io debbo ringraziare, signora Presidente, il senatore Mugnai, per l'intervento di altissimo profilo scientifico che ha svolto nel corso di questa discussione e debbo respingere le censure che, sia pur garbatamente, qualche collega gli ha mosso: il suo è stato l'unico intervento della maggioranza ed è stato un intervento analitico, puntuale, rigoroso, certamente meritevole di quell'apprezzamento Ma, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non si limita soltanto a consentire strumenti di accertamento più profondo nell'ambito del processo. Interviene su alcune vicende di particolare gravità e, rendendosi interprete dell'esigenza avvertita dell'opinione pubblica italiana di trattare con rigore certe condotte che non meritano alcuna considerazione, soprattutto se questa considerazione automaticamente viene consentita dal codice, questo disegno di legge consente che nel giudizio abbreviato, cioè quel giudizio sollecitato da chi ne ha interesse per beneficiare in maniera automatica di una diminuzione di pena, ove mai all'esito delle valutazioni il giudicante, quel magistrato, giudice dell'udienza preliminare, ritenesse che la pena da infliggere debba essere l'ergastolo, questa automatica questa automatica contrazione e riduzione della prova non vi possa essere. Credo che questa rigorosa ipotesi legislativa intercetti un'opinione pubblica diffusa. La gente esige il rigore, e noi le offriamo rigore

quel giudice dell'udienza preliminare che, da solo, con la disponibilità (perché in quel caso egli ha la disponibilità di tutte le carte del processo) degli atti di accusa e difensivi, di accusa e difensivi, analizza, studia, si tormenta sulle carte e, se ritiene che la pena da infliggere debba essere la pena perpetua, la pena più grave, quella dell'ergastolo, allora la sanzione ci sarà, e sarà e sarà grave come deve essere, come il popolo italiano la reclama. E, in nome del popolo italiano, si pronunzierà una sentenza che sia coerente con le aspettative della più vasta opinione pubblica del nostro Paese. Ma questo è il disegno di legge. È la proposta che viene da questa maggioranza: da una parte, un'esigenza di verificare in maniera più puntuale, più ampia, di scandagliare ogni profilo di quegli elementi che poi costituiranno la prova; dall'altra parte, il rigore. Sono due elementi importanti. importanti. Così, signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso tutte queste verifiche e queste ricognizioni, si evita l'altro aspetto del processo, del quale sovente si discute: l'accertamento della verità, da una parte; l'ansia verso l'accertamento della verità, dall'altra. Perché? Per evitare l'errore giudiziario. La storia del mondo è la storia dell'errore giudiziario. Gli errori giudiziari si sono succeduti nel corso dei secoli: da Cristo a Socrate a Dreyfus. La storia è piena di errori giudiziari: momenti importanti della storia del mondo sono stati scanditi e condizionati dall'errore giudiziario. introdotto con questo documento legislativo, nell'auspicio che anche l'altro ramo del Parlamento celermente lo apprezzi e lo approvi, un altro elemento perché sia più difficile sia più difficile che l'errore giudiziario si verifichi, proprio perché il processo deve essere momento dinamico, teso alla verità: due, tre, quattro, cinque testimoni! Ma ben vengano tutti i testimoni che sono necessari per accertare la verità! Mi auguro vivamente che questo disegno di legge possa presto essere legge dello Stato.